Onorevoli senatori, con la legge del 4 maggio 2007, n. 56, è stato istituito il «Giorno della memoria» dedicato alle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice. L'articolo 1 recita: «La Repubblica riconosce il 9 maggio, anniversario dell'uccisione di Aldo Moro, quale "Giorno della memoria", al fine di ricordare tutte le vittime del terrorismo, interno e internazionale, e delle stragi di tale matrice ».

parere favorevole

«La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo ed i relativi emendamenti, esprime, per quanto di competenza, parere di nulla osta sul testo, ad eccezione che sull'articolo 1, comma 3, che, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, dovrebbe essere così riformulata: "*l)* applicazione dei criteri di cui alla lettera anche al fine di valorizzare e incentivare le categorie inferiori e lo sviluppo del settore giovanile e di sostenere gli investimenti ai fini della sicurezza, anche infrastrutturale, degli impianti sportivi;". Esprime infine parere di nulla osta sugli emendamenti».

dei proventi derivanti dalla commercializzazione dei diritti televisivi stessi. Noi proponiamo che i proventi siano così divisi:

1.113. Come ben sanno Governo e relatori, a nome del Gruppo di Alleanza Nazionale abbiamo sostenuto nelle Commissioni riunite alcuni temi, presentando emendamenti poi elaborati,

Vorrei ricordare, tra i vari temi trattati, quello dell'emittenza locale, non solo per quanto riguarda il diritto di cronaca (mentre discutevamo nelle Commissioni riunite, qualche settimana fa, il diritto di cronaca dell'emittenza locale veniva leso in occasione della partita della Nazionale di calcio a Bari), ma anche per la possibilità di acquistare dai *broadcaster* più importanti i diritti delle partite che gli stessi non intendono programmare in palinsesto. Sulla questione delle piattaforme, abbiamo aperto gli occhi a molti colleghi, non solo chiedendo una serie di audizioni importanti (che, come abbiamo sentito anche dai senatori Scalera e Mazzarello, che ringrazio, sono risultate determinanti per migliorare il testo), ma anche presentando una serie di emendamenti e di ordini del giorno

o come la scherma, il canottaggio, il nuoto, la ginnastica, l'atletica: tutte discipline che hanno fatto grande lo sport italiano. L'emendamento 1.113 estende il concetto di mutualità non solo alle infrastrutture sportive e alla sicurezza degli impianti, ma soprattutto a progetti a sostegno di altre discipline sportive. Sono convinto che il calcio professionistico, travolto dalla vicenda delle scommesse, dallo scandalo delle partite truccate, dalla corruzione dilagante, abbia necessità di promuovere diversamente la propria immagine di sport forte, pulito, solidale, aiutando le discipline sportive meno visibili, ma non per questo meno praticate. Il calcio deve promuovere una sorta di mecenatismo verso le discipline più povere. Vorrei ringraziare a tale proposito il sottosegretario Lolli Lolli e i colleghi Mazzarello e Scalera per la sensibilità con cui hanno ascoltato le nostre argomentazioni, giungendo a condividerle ed esprimendo parere favorevole sia sull'ordine del giorno G6 che su questo emendamento. Con l'emendamento 1.113 recheremo un grande beneficio allo sport dilettantistico e apriremo un nuovo rapporto tra un calcio professionistico più attento agli scopi sociali dello sport, più incline alla solidarietà e più onesto sui veri valori dello sport e tutte le altre discipline sportive, più povere economicamente, ma straordinarie per capacità educativa e formativa, non solo delle giovani generazioni.

questa correzione, estremamente limitata, serva soprattutto a meglio specificare il senso della proposta.

si chiede «una procedura trasparente e non discriminatoria» per consentire alle società di realizzare nuovi impianti sportivi

ad intervenire, in sede applicativa (trattandosi di legge delega), con ulteriori e specifici correttivi, al fine di meglio tutelare gli interessi delle emittenti locali, in modo specifico per quanto attiene alla modalità delle trasmissioni in differita degli eventi sportivi a livello locale, tenuto comunque conto dei diversi sfruttamenti dei diritti, senza svilire il valore degli sfruttamenti principali, e della fruizione delle immagini da parte delle emittenti locali che intendano esercitare il diritto di cronaca.

tocca un tema quanto mai attuale: si tratta del raccordo fra produzione di contenuti relativi ad eventi sportivi e loro diffusione con strumenti di comunicazione elettronica. Si pensi, solo per citare un esempio eloquente, alle partite di calcio trasmesse via cavo o via cellulare. Il testo di legge di cui oggi stiamo discutendo contiene proprio princìpi e criteri direttivi per una nuova disciplina relativa alla titolarità ed al mercato dei diritti di trasmissione, alla comunicazione e messa a disposizione al pubblico, in TV e sulle altre reti di comunicazione elettronica, degli eventi sportivi inerenti ai campionati professionistici. La delega intende perseguire due obiettivi fondamentali: garantire l'equilibrio competitivo dei soggetti partecipanti alle competizioni sportive tramite la fondamentale previsione di un nuovo sistema imperniato sulla vendita centralizzata dei diritti televisivi; realizzare un sistema efficace e coerente di misure idonee a garantire la trasparenza e l'efficienza del mercato dei diritti di trasmissione degli eventi sportivi. È bene, dunque, creare norme che perseguano i sopramenzionati obiettivi considerando che, in special modo, gli eventi calcistici costituiscono per gli operatori delle telecomunicazioni un'insostituibile fonte di ricavi. I suddetti eventi sono infatti fattori determinanti ai fini delle dinamiche concorrenziali, ad esempio, nel mercato della raccolta pubblicitaria. Da questo punto di vista, è fondamentale la previsione di una commercializzazione in forma centralizzata dei diritti, con l'esplicita previsione del divieto (divieto importante, contenuto in una mia proposta emendativa assorbita da quella del collega Brutti e approvata nelle Commissioni riunite) di discriminazione tra le piattaforme distributive. Allo stesso scopo concorre la previsione del divieto di acquisire diritti relativi a piattaforme per le quali non si possiede il titolo

accolto dalle Commissioni riunite, di intervenire in sede applicativa prevedendo non solo che gli operatori di comunicazione partecipanti all'acquisizione dei diritti audiovisivi sportivi siano in possesso del titolo abilitativo, ma che effettivamente lo esercitino. Gli eventi calcistici e di altri sport (quali la pallacanestro, il ciclismo, il motociclismo, il pugilato, il golf) possono essere sicuramente considerati mezzi di forte impatto per lo sviluppo e l'affermazione delle cosiddette piattaforme emergenti emergenti (digitale satellitare, digitale terrestre, cavo, UMTS, Internet o banda larga, analogico terrestre in chiaro). Non a caso, infatti, una speciale disciplina dovrà essere emanata proprio per le piattaforme emergenti, così come previsto dal criterio contenuto alla lettera *g)* del comma 3. Tale lettera è stata opportunamente modificata, con l'accoglimento nelle Commissioni riunite di parte di un emendamento a mia firma, sostenuto anche da altri colleghi. La suddetta modifica all'originario testo consiste nell'introduzione della previsione esplicita di misure di sostegno della concorrenza da introdurre nei decreti delegati. Concludendo, annuncio, a nome dei Popolari-Udeur, il voto favorevole sul provvedimento in esame.

considerazioni. L'istituto della delega su una materia così vitale per il mondo dell'informazione non è accettabile né condivisibile. Quindi, espressa tutta la contrarietà al ricorso a questo istituto per trattare un tema così delicato, mi auguro che il Governo metta quanto prima

la gestione di una materia che, tra l'altro, è in continua evoluzione anche per il moltiplicarsi delle società sportive, degli eventi sportivi, delle emittenti televisive, quindi degli attori di questa scena. Mi sembra utile ricordare i princìpi del parere espresso, che si apre proprio con il rifiuto della delega come strumento per risolvere questi problemi, ma con qualche commento favorevole su taluni aspetti che il disegno di legge propone: per esempio, riguardo le norme sulla commercializzazione in forma centralizzata, che dovranno garantire forme di partecipazione di tutte le piattaforme sia per evitare distorsioni sempre dannose del mercato, sia soprattutto per garantire i diritti delle emittenti locali - la parte più debole su questo mercato affinché possano competere con pari opportunità con le emittenti più forti nella distribuzione degli eventi sportivi. C'è ancora l'esigenza di tutelare maggiormente soprattutto le emittenti locali laddove le grandi emittenti non manifestino interesse a gestire l'evento sportivo. In questo senso, mi sembra inopportuna la misura di vietare le sublicenze, vale a dire la possibilità, a fronte del disinteresse dell'emittente che ha la titolarità dell'evento, di cedere la possibilità di rappresentarlo ad emittenti locali, che viceversa hanno tutto l'interesse a farlo. Eviteremmo in questo modo anche il pericolo di fastidiose discriminazioni nei confronti di organizzatori di eventi sportivi, i quali, dichiarati non interessanti dalle grandi emittenti, non avrebbero un'adeguata copertura televisiva. C'è poi un importante aspetto nella distribuzione delle risorse: non bisogna dimenticare l'esigenza di garantire una certa mutualità tra le diverse discipline sportive per fare in modo che le più ricche, le più forti, e così anche le società, sostengano lo sport di base, lo sport dilettantistico, vale a dire quelle forme di attività sportiva diretta dei cittadini che altrimenti non avrebbero supporto. La nota che correda il parere della 10a Commissione si chiude con un accenno al diritto di cronaca, una formalità formalità che si è inserita negli ultimissimi anni, da quando il monopolio della RAI è stato attaccato e intaccato in taluni settori dall'attività delle emittenti private.

esempio, rifiuta il ricorso a quella che veniva definita un tempo la criptazione per trasmissioni ritenute di interesse generale e sociale. Penso in modo particolare ai grandi eventi del calcio, ai mondiali, alle partite delle nazionali, che in certi Paesi venivano criptate perché non esistevano contratti chiari. Per Per quanto riguarda le sub-licenze, vi è una raccomandazione da rivolgere al Governo: esse costituirebbero un elemento di giustizia e di parificazione per le emittenti private locali, anchele più piccole, laddove intervengano accordi preliminari - come sempre accade - tra gli organizzatori di eventi e chi vince il bando di concorso. Succede poi nel tempo poi nel tempo che chi acquisisce il diritto scopra che non lo può esercitare, o per un interesse di carattere tecnico-giornalistico o magari per mancanza di risorse. In quel modo l'organizzatore dell'evento viene privato della possibilità di vedere la diffusione dell'evento attraverso le forme televisive. In questo caso, non sarebbe assolutamente scandaloso né contro le regole se

attinente un livello minimo garantito di qualità della trasmissione, in quanto, se vi sono vincoli per l'acquisizione di un diritto, non si può poi svendere sul libero mercato a chiunque possa esercitarlo, magari senza avere la possibilità di portarlo avanti con livelli e *standard* di qualità. Infine vorrei tornare sul tema del diritto di cronaca. In tale campo il Governo deve intervenire in maniera chiara, soprattutto di fronte al moltiplicarsi delle emittenti televisive. Ricordo con molta

Fu per tutti gli operatori della RAI, in quel momento, uno *shock* in quanto quel tipo di servizio era considerato una cosa di famiglia. In quel momento, scattò il difficile e delicato esercizio del diritto di cronaca. La RAI doveva dare ai suoi utenti, semplicemente, tre minuti al giorno. Non ci si può affidare a un rimedio empirico e incerto come questo e lascio al Governo, in chiusura, la raccomandazione

Presidente, onorevoli colleghi, rappresentanti del Governo, crediamo che l'approvazione della delega sia un passaggio importante per guardare con maggior speranza al futuro dello sport, e del calcio in particolare. Durante i lavori relativi a questo provvedimento, diversi oratori nei loro interventi si sono interrogati sui motivi della crisi che vive il calcio nel nostro Paese, crisi innanzitutto morale, che è indipendente dai risultati sportivi. Non si può fare finta che gli eventi che dal maggio del 2006 si sono succeduti e hanno portato al commissariamento della Federazione italiana giuoco calcio siano stati superati con una bacchetta magica. Certo, il ruolo del commissario è stato importante per imprimere una svolta nei costumi e nei comportamenti del panorama calcistico, tanto più di fronte al riesplodere della violenza, ma resta ancora molto da fare. Ci riferiamo a questa situazione perché siamo convinti che questi siano anche gli effetti di un modello deteriore, che ha avuto nella concorrenza, non sportiva ma economica, introdotta con la contrattazione individuale dei diritti televisivi uno dei suoi motivi principali. Il ritorno alla contrattazione collettiva è una buona strada per affermare un principio di fondo che, speriamo, indirizzi le nostre scelte future: l'autonomia del mondo sportivo non si ottiene senza una mutualità, senza forme di solidarietà, senza che ciascuno, per il suo ruolo, sia chiamato a chiare assunzioni di responsabilità. Se una società o una federazione travalica il principio di mutualità diventa allora complicato assicurare l'autonomia. Se il calcio, o qualunque altro sport professionistico, è solo mercato e profitto, è difficile esigere uno *status* diverso da quello garantito a tutte le altre imprese che operano nel Paese. È per questo che tanto noi quanto altri Gruppi di maggioranza e opposizione abbiamo sollecitato che una parte delle risorse andasse ad assicurare la sicurezza negli eventi sportivi: queste sono le assunzioni di responsabilità che, di fronte al fenomeno drammatico della violenza, ci aspettiamo e auspichiamo. La destinazione di una quota della mutualità al fine di incentivare gli investimenti nell'impiantistica sportiva, oggi tema centrale nel progetto di riforma dello sport che il Governo sta intelligentemente portando avanti, e la destinazione di una quota ai fini di finanziare, attraverso fondazioni create *ad hoc* dalla Lega calcio, progetti sia nel sociale che nell'ambito della scuola e dell'università, sono segni chiari di una strategia seria e pensata. Esistono caratteri precipui dell'attività sportiva che sono eminentemente sociali e non economici. Non si tratta di demonizzare il mercato, ma di porre a tema la questione di un giusto equilibrio tra effetti sociali dell'attività sportiva e conseguenze economiche, come posto chiaramente nella Dichiarazione di Nizza che il provvedimento richiama. Anche per questo ci sembra che questo provvedimento inverta la tendenza, e speriamo che accompagni una vera e propria riforma del nostro mondo calcistico. L'etica richiamata dal neopresidente della FIGC Abete, in occasione del suo insediamento, è un buon auspicio, e questo primo provvedimento è uno strumento utile per garantire trasparenza allo sport. Forse le future candidature italiane ad eventi di portata internazionale si potranno giovare di un sistema più trasparente e meno subalterno alle sole logiche di mercato. Questo provvedimento, allora, può essere un importante momento di svolta per il calcio, ma lo può essere anche per rilanciare le nuove tecnologie nel nostro Paese; è evidente come il calcio sia il contenuto trainante delle nuove potenzialità che ci sono offerte dallo sviluppo della tecnica: dal digitale terrestre ad Internet assistiamo ad un fiorire di nuove opportunità, anche imprenditoriali e occupazionali. Perché questa innovazione abbia seguito è necessario che gli operatori consolidati nei vecchi *media*, come la televisione analogica, non cerchino di sfruttare la propria posizione dominante, perché questo sarebbe un freno grave allo sviluppo complessivo del Paese. Anche in questo caso credo che abbiamo svolto un buon lavoro, migliorando quella che era già una buona base di partenza. La scelta di garantire la libera concorrenza nel mercato dei diritti di trasmissione, senza discriminazione tra le piattaforme distributive, l'obbligo di trasmissione, rimuovendo la possibilità che soggetti dominanti acquisissero i diritti per ritirarli dal mercato, l'opportunità delle vendite in modo trasparente, non discriminatorio e a prezzi equi tra le diverse piattaforme consentono di promuovere un mercato delle telecomunicazioni davvero concorrenziale e aperto. Le vicende a cui abbiamo assistito relativamente al digitale terrestre e, prima ancora, ai servizi via satellite hanno dimostrato come sia proprio lo sport il contenuto che consente alle diverse piattaforme tecnologiche di decollare, e con questo provvedimento forse riusciremo a porre un primo tassello per liberalizzare un mercato, quello delle telecomunicazioni, che nel nostro Paese è attardato da un'organizzazione vecchia e in affanno, che ruota ancora intorno al duopolio televisivo. Finalmente si riconosce chiaramente che i diritti di trasmissione sorgono *ab origine*, in capo agli allestitori dello spettacolo sportivo, cioè ai club e alla Lega calcio, in modo che il sistema dei diritti sia dotato di idonea protezione contro determinati fenomeni di natura illecita: ad esempio, contro quello della captazione illecita e della illecita immissione in rete delle immagini delle partite, fenomeno sempre più crescente (si veda, da ultimo, la causa intentata alcuni giorni fa dalla *Premier* *League* contro *YouTube*). Ma il tema del diritto d'autore e del diritto di cronaca necessiteranno di un lavoro puntuale del Governo, per trovare il giusto equilibrio tra la vendita del diritto e la disponibilità degli eventi come fattore sociale e identitario. Per tutti questi motivi, laddove la legge delega, sulla base di un nostro emendamento recepito in Commissione, richiama l'«alveo della tutela dei diritti riconosciuti dall'ordinamento ai diritti di trasmissione», si vuole far sì che il Governo, nel momento dell'attuazione, predisponga una disciplina specifica e concreta, che dia protezione e accessibilità ai diritti audiovisivi sportivi. Se quindi lo sport può favorire la creazione di un mercato delle telecomunicazioni più libero, non bisogna però però dimenticare il valore sociale della pratica sportiva. Le scelte di salvaguardia dell'emittenza locale, anche con una specifica disciplina per i diritti secondari, vanno proprio in questa direzione. Le scelte contenute in questo provvedimento consentono quindi di ridare slancio al processo di riforma che sta investendo il mondo del calcio: insieme al decreto contro la violenza negli stadi, quello di oggi è un passaggio importante per riaffermare trasparenza e autonomia del pallone. Restano aperti, rispetto alle sfide che ci eravamo dati, altri due importanti tasselli, cioè la valorizzazione dell'attività sportiva tra i giovani e nelle scuole e il grande tema della proprietà degli stadi in capo alle società sportive. Proprio sui giovani occorre porre la massima attenzione: bene il provvedimento oggi all'esame, che mette l'accento sul problema degli investimenti sui vivai; bene il Ministero per le politiche giovanili e per le attività sportive, che in questi mesi ha posto in essere iniziative, anche a livello locale, come nel caso ultimo della Campania, che vede lo sport come sistema per la crescita e lo sviluppo del mondo giovanile; bene qualsiasi futura iniziativa parlamentare che, di concerto con le istituzioni sportive e nel rispetto della loro autonomia, possa risolvere i problemi connessi allo svolgimento delle attività sportive, non solo professionistiche, che vedono coinvolti soprattutto i ragazzi nella fase adolescenziale. Siamo quindi ad un importante provvedimento complessivo sul calcio e sullo sport nel suo complesso. Non vorremmo, infatti, che la preminenza economica che il calcio ricopre mettesse in ombra il valore complessivo che questo intervento ha per tutto il sistema sportivo: non solo si risolve una questione ormai annosa, quella del calcio, ma si consegna al Governo la responsabilità di definire una normativa moderna, capace di promuovere la totalità degli eventi sportivi professionistici a squadre. Cogliamo qui una grande opportunità per il rilancio di quegli sport che, se sono meno visibili nelle cronache, sono seguiti e praticati da migliaia di cittadini e rispetto ai quali la trasmissione sulle diverse piattaforme può essere una grandissima opportunità di visibilità e di rafforzamento. Lo strumento della delega, aspramente criticato da alcuni, probabilmente in un contesto come questo si rivela il più efficace: da un lato, siamo di fronte a cambiamenti tecnologici estremamente rapidi e incisivi, e i decreti e le eventuali correzioni consentono di affrontare questa evoluzione con la necessaria flessibilità; dall'altro, la presenza di soggetti importanti non solo economicamente ma anche dal punto di vista sociale richiede, nei puntuali limiti disposti dalla delega, un'azione di coordinamento e concertazione che sia capace di rilanciare il sistema sportivo italiano. Oggi quindi licenziamo un provvedimento che può consentire tre importanti risultati. Il primo è la grande opportunità per la moralizzazione del nostro calcio, e perché dopo le bufere degli ultimi mesi il gesto sportivo sul campo torni davvero protagonista, e non siano le intercettazioni e le corruzioni a riempire il dibattito nazionale. Il secondo è la promozione del complesso dello sport nazionale, con un ruolo non più marginale per i grandi eventi a squadre. Il terzo Il terzo è la nascita di un sistema delle telecomunicazioni più aperto, dove la concorrenza non sia solo tra i soliti noti e l'innovazione non sia guardata con sospetto.

Signor Presidente, onorevoli colleghi, il voto che ci troviamo oggi ad esprimere è il voto su un provvedimento che costruirà un nuovo scenario nel settore radiotelevisivo e che purtroppo rischia di non cogliere nel segno e quindi di non raggiungere l'obiettivo sperato. Anche la Lega Nord insegue l'equilibrio competitivo, condivide la necessità di un provvedimento che limiti il diritto soggettivo alla vendita dei diritti TV e reintroduca la contrattazione congiunta da parte della Lega professionisti, ma non può appoggiare un disegno di legge come quello oggi in esame in cui, utilizzando l'inadeguato strumento della delega legislativa, non sono specificati i diversi criteri di ripartizione dei proventi; non viene destinata una quota fissa alla crescita del movimento di base; non si prevede chiaramente la condizione di libero mercato per la vendita su una singola piattaforma con divieto di sub-licenza. Sono tutti aspetti fondamentali, che avrebbero dovuto indurre questo Governo ad affrontare l'esame del provvedimento con maggiore cautela, quella stessa cautela che aveva peraltro contraddistinto i vostri colleghi del 1999 quando, con un decreto‑legge, era stata posta l'attenzione su un settore allora nascente, la televisione digitale e satellitare. Allora, intuita la posta in gioco, si imponeva una rigida suddivisione dei diritti tra i due concorrenti. Così non è stato ora. Abbiamo cercato un dialogo per dare il nostro contributo al fine di migliorare il provvedimento presentando emendamenti contenenti misure per il movimento di base, per l'impiantistica, per i giovani, per la formazione tecnico‑professionale dei formatori, ma voi avete preferito ignorare i nostri suggerimenti. Le nostre proposte emendative, partendo dal presupposto che lo sport si fonda su valori sociali, educativi e culturali, erano volte a far sì che i proventi incassati dalle federazioni per la contrattazione collettiva dei diritti televisivi venissero destinati in modo specifico, con quote ben definite, al movimento di base. Pensiamo infatti che le associazioni sportive hanno il dovere di promuovere lo sport che rappresentano attraverso i vivai, l'attività giovanile, l'inclusione sociale dei giovani sportivi e non solo. Tutto questo non è presente nel provvedimento, è abbozzato nella relazione e se ne parla genericamente nell'articolato, ma non viene affrontato in termini concreti. Nel momento in cui nel provvedimento si stabilisce come ripartire le importanti ed uniche risorse su cui il mondo sportivo può contare, ossia quelle provenienti dai diritti televisivi, ci si dimentica di dare direttive precise, di definire le quote di riferimento per le federazioni o per le leghe da destinare alla missione che esse hanno. Una buona legge sul riordino dei diritti televisivi, in analogia con quanto già previsto in altri Paesi europei, non può non prevedere misure specifiche per la valorizzazione di vivai giovanili nello sport. Nella redistribuzione proposta in questo disegno di legge, invece, non viene preso in considerazione l'investimento di ciascun partecipante nell'attività del vivaio, punto fondamentale per la Lega Nord. Per quanto riguarda la mutualità interna ai singoli campionati, abbiamo proposto una redistribuzione delle risorse in base alla rilevazione dei minuti complessivamente giocati in prima squadra dai giovani giocatori di cittadinanza italiana cresciuti nei vivai, sulla base di quanto prevede il regolamento utilizzato dalla Lega calcio, ma anche questo suggerimento è caduto nel vuoto. Non possiamo allora accontentarci del testo così come è stato discusso oggi, quando si parla di una quota non quantificata da destinare alla mutualità generale del sistema: la Lega Nord ritiene una questione dirimente definire questa quota al 10 Lo sport deve tornare ad essere un motore sociale positivo e deve recuperare la sua funzione educativa e culturale. Per far sì che ciò accada è fondamentale che le ingenti risorse che è possibile recuperare attraverso la vendita collettiva vengano ben utilizzate; così purtroppo non è stato in passato. L'abbiamo appreso dalle numerose indagini svolte dal Parlamento e dall'autorità. Il secondo tema su cui vorrei richiamare l'attenzione di quest'Aula è che il provvedimento è lacunoso anche per quanto riguarda l'aspetto televisivo. Noi tutti sappiamo che la trasmissione degli eventi sportivi, e in particolare del calcio, ha assunto un ruolo strategico per l'economia del settore, superando nel fatturato prodotti d'intrattenimento e cinema. Le televisioni a pagamento, a differenza delle TV generaliste, che dipendono dalle inserzioni pubblicitarie, sono strettamente legate alle preferenze e ai consumi degli abbonati: la vendita dei diritti delle partite di calcio oggi addirittura copre quote di tre quarti del fatturato. I contenuti calcistici costituiscono, tanto per gli operatori televisivi in chiaro quanto per gli operatori televisivi a pagamento, un'importante fonte di ricavi pubblicitari e rappresentano, anche in prospettiva, fattori determinanti ai fini della definizione delle dinamiche concorrenziali nel settore televisivo, ed in particolare nel mercato della raccolta pubblicitaria sul mezzo televisivo. Ne consegue che la vendita dei diritti, combinata alla portata dell'esclusiva, ha effetti significativi sulla struttura dei mercati, in quanto può favorire la concentrazione dei *media* ed ostacolare la concorrenza fra le emittenti. I diritti TV degli eventi sportivi, e soprattutto calcistici, determinano una particolare immagine di marchio per il canale che li trasmette e consentono alle emittenti di raggiungere un particolare pubblico, non altrimenti raggiungibile con altri programmi. Nei canali a pagamento, il calcio è la principale forza trainante per la vendita di abbonamenti, mentre nella TV non a pagamento il calcio attrae una particolare fascia di pubblico e, di conseguenza, inserzionisti pubblicitari che non sarebbero attirati da altri programmi. Parlo del calcio perché, diversamente da altri sport, il calcio consente, alle emittenti che ne acquisiscono i diritti, di ottenere cifre elevate di spettatori su base regolare, prolungata e continua, con i conseguenti benefìci in termini di introiti pubblicitari o abbonati ai servizi a pagamento, al punto che il prezzo degli intermezzi pubblicitari durante la trasmissione del calcio è maggiore del 10-50 per cento rispetto al miglior prezzo praticato. Sebbene vi siano eventi di campionati di altri sport e sebbene tali sport siano in grado di produrre *audience* maggiori, non raggiungono la stessa costanza di numero di spettatori del calcio. Si può quindi affermare, con decisione e chiarezza, che il contenuto calcistico è un fattore determinante ai fini della definizione delle dinamiche concorrenziali nel settore televisivo. Abbiamo evidenziato come sia necessario introdurre specifici correttivi in un mercato rilevante come quello dell'acquisizione dei diritti di trasmissione delle competizioni sportive, e in particolare calcistiche, che con questo disegno di legge stiamo determinando quali saranno in futuro i soggetti che, rispetto ad altri, potranno avvantaggiarsi nell'acquisizione di quei diritti. È chiaro quindi, date le premesse, che la possibilità di trattare su una singola piattaforma di gara significherebbe che, laddove non vi saranno *competitor* (per quanto riguarda la TV a pagamento così non è), ci troveremo ad avere un solo concorrente. Un po' di buonsenso porta a pensare che questo risulta in conflitto con qualsiasi idea di gara, di libero mercato e, comunque, è molto lontano dall'idea, formulata dallo stesso Governo, di aumentare il volume dei ricavi a favore dello sport. Dopo tutte queste considerazioni, signor Presidente, il nostro parere è che non c'è nulla di innovativo in questo provvedimento: non ci sono risorse per i giovani, nessuna misura per lo sport dilettantistico, una pessima mutualità interna, ed è fallita anche quella condizione fondamentale di rispetto delle dinamiche concorrenziali. Pertanto, il voto della Lega Nord non può che essere contrario a questo provvedimento. Signor Presidente, colleghi senatori, rappresentanti del Governo, il disegno di legge delega che ci apprestiamo a votare è entrato, credo non volendolo, nell'attualità della vita sportiva del nostro Paese. Infatti, quando l'*iter* di questo provvedimento è stato avviato alla Camera dei deputati, sconvolgenti fatti di cronaca nera erano accaduti e purtroppo altri ne sarebbero seguiti prima, durante e dopo determinati eventi sportivi. La legge in questione, quindi, ha risentito di questo clima, ma credo che la cosa non sia stata per nulla negativa, anzi. Infatti, la risposta che il testo ha dato alle esigenze del momento non è stata né emotiva né demagogica. Si è ragionato con serenità, respingendo ogni tentativo di criminalizzare lo sport, il calcio in modo particolare, sia in relazione alle vicende di Calciopoli, sia per gli squallidi e drammatici casi di criminalità, nei quali i soliti, pochi delinquenti hanno macchiato lo sport più amato e seguito dagli italiani. Sarebbe stato comunque un errore colpire le società attraverso la disciplina dei diritti di trasmissione degli eventi sportivi per il semplice fatto che questi non rappresentano un beneficio solamente per il calcio ma per tutte le società sportive. Un clima pesante e per molti aspetti negativo intorno allo sport ha prodotto invece, a nostro giudizio, un buon testo di legge perché ha messo in modo forte e consapevole un nuovo senso di responsabilità che, partendo dalla più alta istituzione del Paese, il Parlamento, ha avviato una serie di nuovi comportamenti ed una nuova cultura, che speriamo riuscirà ad invertire una tendenza che ha prodotto un clima di sfiducia e di giudizi decisamente negativi da parte della pubblica opinione. Tutti, quindi, dalle società sportive alle tifoserie, agli stessi sportivi, in particolare i professionisti, sono responsabilizzati verso comportamenti più virtuosi, pena un discredito che finirebbe per danneggiare in modo irreparabile l'immagine dello sport nel nostro Paese. Questo non possiamo permettercelo, anche perché lo sport è oggi la prima occasione di aggregazione per i nostri ragazzi e per i nostri giovani; per molti di loro l'unica occasione per passare in modo sano, pulito e costruttivo il tempo libero dal lavoro e dagli impegni scolastici. L'UDC ritiene, per quello che è di propria e stretta competenza, che il disegno di legge n. 1269 risponde a queste urgentissime esigenze di natura sociale. Vi sono alcuni aspetti qualificanti della legge che vorrei mettere in risalto, per motivare il voto positivo del Gruppo dell'UDC. Il primo riguarda l'emendamento, da noi presentato, che sostituisce integralmente la lettera *c)* del terzo comma dell'articolo 1. Questo prevedeva la disciplina della commercializzazione in forma centralizzata dei diritti sul mercato nazionale per singola piattaforma. Tale disposizione avrebbe inevitabilmente attribuito posizioni dominanti a singoli operatori, dove la divisione appunto per singola piattaforma finiva per assicurare in modo quasi automatico ad un singolo operatore determinate trasmissioni di eventi sportivi. Su questo specifico punto i nostri colleghi della Camera hanno cercato di fare controproposte, che non sono state a suo tempo accolte. Alla fine dell'*iter*, l'UDC si asteneva sul testo, che riteneva per il resto sostanzialmente positivo. In sede di Commissioni riunite 7a e 8a del Senato, l'UDC ripresentava l'emendamento che sostituiva integralmente questa parte del testo. L'emendamento è stata accolto e questo fa mutare il nostro convincimento: dall'astensione al voto favorevole. Questo comportamento rientra in quell'atteggiamento più generale di opposizione responsabile che caratterizza le nostre scelte politiche e che ci porta in sede parlamentare a contribuire, a volte in modo decisivo come in questo caso, all'approvazione di buoni testi di legge, equilibrati e condivisibili. La modifica che abbiamo apportato al comma 3 cambia radicalmente la disciplina della commercializzazione in forma centralizzata dei diritti, perché tiene conto del veloce mutamento della tecnologia nel settore delle comunicazioni, contempla procedure di regolamentazione e vigilanza da parte dell'Autorità per le garanzie delle comunicazioni e dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato che prima non erano previste e prevede che le stesse Autorità possano concedere limitate deroghe finalizzate ad assicurare pari diritti agli operatori della comunicazione ed il non formarsi di posizioni dominanti, sicché siano meglio tutelati gli interessi del soggetto preposto all'organizzazione della competizione sportiva. Su questa stessa linea, è stata non di poco conto la modifica, alla lettera *h)*, della previsione della «durata ragionevole dei contratti aventi ad oggetto lo sfruttamento dei prodotti audiovisivi». Quel «ragionevole» appariva decisamente inadeguato e troppo indefinito. Saggia è stata pertanto la decisione del relatore e del Governo Governo di accogliere gli emendamenti, fra cui il nostro, che prevedevano una durata dei contratti non superiore ai tre anni, allo scopo di garantire l'ingresso nel mercato di nuovi operatori e di evitare, appunto, la creazione di posizioni dominanti. Allo stesso modo, è rigidamente garantito il diritto di cronaca per tutti gli operatori del settore, così come si cerca di salvaguardare le esigenze dell'emittenza locale, grazie al testo approvato dalle Commissioni riunite, nella lettera *b)* del comma 2. Questo garantisce la copertura per ogni tipo di evento sportivo ed inserisce piccole radio e TV locali nel grande circuito delle trasmissioni sportive. Queste, in sintesi, le regole che la disciplina della commercializzazione dei diritti prevede: nessun vincolo di assegnazione per singola piattaforma; ampia possibilità di concorrenza a garanzia di tutti gli operatori della comunicazione, ma anche evidenti vantaggi di maggiori introiti economici per le società sportive (grazie appunto alla maggiore concorrenza); cogenti norme a garanzia del diritto di cronaca; limite oggettivo al formarsi di posizioni dominanti; largo favore assegnato alle emittenti locali. Mi permetto di richiamare il Governo al riguardo del parere della 14a Commissione, laddove, pur esprimendo parere favorevole, essa ritiene necessario prevedere che la regolamentazione che sarà predisposta dal Governo in attuazione della delega sia sottoposta all'attenzione della Commissione europea (ai sensi dell'articolo 81, paragrafo 3), perché 3), perché ci sia un'attenta valutazione per l'accesso anche delle piccole emittenti, così che sia effettivamente garantita la parità di trattamento di tutti gli operatori della comunicazione. Infine, crediamo sia stata decisiva l'impostazione data dalla lettera *i)*, dove si stabilisce che una quota prevalente delle risorse sia ripartita in parti uguali a tutte le società sportive. Quel «prevalente», intorno al quale si è molto discusso, non è un numero vincolante per il soggetto titolare dei diritti (quindi ne rispetta l'autonomia e la libertà), ma è un'indicazione forte, che si accompagna a quanto previsto nei punti successivi per la destinazione di una quota delle risorse ai fini di mutualità generale del sistema. Anche qui, dunque, possiamo indicare alcuni punti di riferimento chiari. Primo: equa distribuzione della parte prevalente delle risorse. Secondo: mutualità generale del sistema. Terzo: valorizzazione del settore giovanile e delle categorie inferiori. Quarto: investimenti per la sicurezza degli impianti. Altri argomenti, questi, più che sufficienti per motivare il nostro voto favorevole ad una legge alla cui formazione l'UDC ha contribuito in modo significativo. finestra"). Vorrei segnalare all'Aula la presenza nelle tribune di una delegazione della Facoltà di scienze politiche dell'Università di Genova, capitanata dal collega Armaroli, cui rivolgo un saluto e gli auguri di buon lavoro.

stiamo portando a conclusione il dibattito su un provvedimento legislativo particolarmente complesso, sia per i contenuti, sia per il contesto in cui esso si inserisce.

nella vita dello sport più amato e seguito in Italia, il calcio, in una stagione difficile e di crisi, in un'epoca in cui quel grumo di passione popolare per la squadra, di professionalità e di spirito sportivo, collettivo e solidale, di legame fra pratica sportiva nel territorio e realtà calcistica professionistica locale si sono distorti e vengono attraversati da decadenza dei comportamenti e degenerazione dei fini. Tutto ciò è causato dalla totale messa sul mercato della competizione sportiva, della squadra, del risultato, dell'atleta e della diretta. La biografia, per certi aspetti drammatica e contraddittoria, del grande atleta Maradona è un po' la metafora del calcio, non solo italiano, nell'epoca della globalizzazione neoliberista. pertanto in un contesto in fibrillazione. Abbiamo alle spalle gli episodi violenti negli stadi italiani, con una vita spezzata e anche l'intervento legislativo urgente che abbiamo votato per porvi rimedio, che ha tutte le caratteristiche e anche i limiti dei provvedimenti emergenziali, e precedentemente lo scandalo di Calciopoli, per cui si sono mossi la giustizia sportiva, la magistratura ed anche il Parlamento con ben due indagini conoscitive alla Camera, una del 2004 e un'altra ancora in corso. Rimuovere e analizzare le cause della crisi è quindi necessario, ma non è né semplice né banale. Questo può farlo innanzitutto la società dello sport e del calcio, nella sua autonoma volontà di riforma e di autogoverno, ma anche la politica e, in particolare, il Parlamento nella sua funzione legislativa. tratta di un'ingerenza indebita: lo sport è un valore sociale, non un fatto privato. Uno dei fattori di tale crisi, accertata da più fonti, è lo squilibrio fra le squadre, tre grandi squadre del Nord e due di Roma, irraggiungibili nei proventi ottenuti dalla vendita individuale dei diritti televisivi, che rappresentano la maggior parte delle entrate di una squadra. modo, le squadre più ricche si sono quotate in Borsa, e il valore delle loro quote societarie, il profitto a Piazza Affari è diventato molto più importante del risultato sportivo. nell'ubriacatura neoliberista di destra, che ha attraversato anche il centro-sinistra, hanno perfino pensato a un certo punto di intervenire con provvedimenti eccezionali a favore delle società indebitate. Il mercato insomma non si è rivelato amico e alleato dello sport, ma fattore di una sua decadenza. Altre sono le regole che lo devono attraversare per recuperare la sua funzione sociale. Da tale assunto parte questo provvedimento legislativo, che incrocia i temi dello sport e della sua funzione sociale a quelli delle regole del mercato e della comunicazione. Tale intreccio è complicato e tale complessità è anche significata dalla modalità del dibattito istruttorio, che ha visto la 7ª e l'8ª Commissione lavorare costantemente in modo congiunto e interdisciplinare, con una prevalenza però

il nucleo forte e ordinatore della legge fosse esclusivamente la questione del mercato della comunicazione. Vorrei che qui si capovolgessero le priorità. Penso che il senso del cambiamento che introduciamo, la discontinuità con il passato sta innanzitutto nel rimettere al centro le finalità dello sport, quelle ricordate dalla Dichiarazione di Nizza del dicembre 2000, dove lo sport viene definito «un'attività umana, che si fonda sui valori sociali, educativi e culturali essenziali» e ancora «un fattore di inserimento, di partecipazione alla vita sociale, di tolleranza, di accettazione delle differenze e di rispetto delle regole», ossia un fattore di rimozione delle disuguaglianze. Lo sport può costituire per le squadre fonte di reddito e attività economica solo dentro questi limiti, quelli che la legge chiama giustamente princìpi (e sono princìpi sovraordinatori), da cui tutto discende di cui vale la pena ricordare il primo, cioè «il carattere sociale dell'attività sportiva quale strumento di miglioramento della qualità della vita e mezzo di educazione e sviluppo sociale». Il disegno di legge n. 1269 interviene sulla distribuzione dei profitti di questa attività economica derivante dalla vendita dei diritti televisivi (ciò è possibile modificando radicalmente e in modo sostitutivo il decreto-legge n. 15 del 1999, convertito nella legge n. quindi, la titolarità dei diritti di trasmissione è del soggetto organizzatore; si introduce, poi, il concetto di contitolarità e si stabilisce che la vendita dei diritti è centralizzata e che la distribuzione delle risorse viene effettuata con criteri mutualistici e solidaristici. Per la centralizzazione della vendita, ci uniformiamo alla prassi di altri Paesi europei (come la Francia, l'Inghilterra e la Germania), che hanno una grande tradizione calcistica, consolidata e di qualità. insomma, anche in linea con i recenti orientamenti europei in materia disport, elaborati nel rapporto indipendente sul calcio europeo del 2006. La contitolarità fra soggetto organizzatore e singola società calcistica avvantaggia, di fatto, le cosiddette società minori, perché la vendita centralizzata è un volano per l'acquisizione delle risorse e restituisce valore anche ai piccoli eventi sportivi. Proprio questa concentrazione delle risorse permette una redistribuzione che coniuga due criteri: in primo luogo, l'equa ripartizione fra i soggetti partecipanti alla competizione sportiva, per assicurarne l'equilibrio competitivo (equa ripartizione che tiene conto del bacino di utenza e anche dei risultati della squadra); in secondo luogo, la destinazione di una quota con finalità mutualistica e di sistema, indirizzata alla valorizzazione dello sport giovanile ed alle categorie inferiori (auspichiamo e ci batteremo affinché questa quota sia significativa). È importante che si invitino le Leghe a elaborare regole e precisare la ripartizione delle risorse secondo i criteri indicati; ciò costituisce un atto concreto di fiducia nell'autogoverno del mondo sportivo. E, per finire, questa legge garantisce anche la regolarità del mercato, le pari opportunità per tutti gli operatori della comunicazione in possesso del titolo abilitativo e la lealtà della concorrenza, tenendo conto sia della rapidissima evoluzione tecnologica del settore sia della problematica relativa alle cosiddette piattaforme emergenti, cioè le posizioni di chi parte in evidente svantaggio (perché soggetti o situazioni disuguali richiedono diritti asimmetrici). voteremo con convinzione a favore di questa legge, come un primo passo per il riordino del sistema calcistico, attenti, in modo particolare, alla fase di transizione che si prospetta difficile e complicata.

senatori relatori, io - che sono un inguaribile ottimista - credo che il Senato abbia svolto oggi (e non solo oggi, ma anche nei giorni scorsi) un lavoro di qualità relativamente al provvedimento

Del resto, trattare compiutamente le complesse questioni attinenti al mondo dello sport non è facile come girare su un pullman scoperto per le vie di Roma, tra i calciatori campioni del mondo, dispensando baci come se si fosse segnato l'ultimo gol.

abbia fatto veramente bene ad affidare le sorti di questo provvedimento ai sottosegretari Lolli e Vimercati, evitando di calcare le scene delle competenti Commissioni al Senato. Credo che ciò abbia agevolato il dibattito. Certamente, la sua presenza qui oggi, quanto meno al momento del voto finale, sarebbe stata cosa gradita.

Noi ci asterremo non tanto perché qualche passaggio non lo riteniamo del tutto convincente, ma perché con lo strumento della legge delega il Governo ha strozzato il dibattito parlamentare, che ciò nonostante si è sviluppato in modo sereno, interessante e competente in Senato. Questo significa che il Parlamento avrebbe potuto anche partorire, lo dico ai colleghi del centro-sinistra in modo particolare, un testo più completo, più coraggioso, più denso anche di significato politico. Ma in quest'Aula regna il terrore della discussione, c'è l'idiosincrasia per il voto elettronico. Attribuite al voto sugli emendamenti e sui provvedimenti un significato decisamente superiore rispetto a quello di un sano e corretto confronto politico.

Non avremo tante altre occasioni di confrontarci sulla questione educativa e pedagogica che anima lo sport, fuori da ogni retorica, sui problemi che le federazioni sportive incontrano ad entrare nel mondo della scuola, così disattenta verso la pratica delle discipline sportive, sulle difficoltà economiche di molte federazioni e, più in generale, del CONI. Credo che il Parlamento abbia il diritto e - aggiungo - il dovere di entrare in queste materie. Certo, ci siamo occupati di violenza negli stadi, ma solo dopo avere accusato l'ennesimo lutto tra le forze dell'ordine. Ci siamo occupati di infrastrutture e investimenti, salvo poi vedere naufragare la nostra candidatura per gli Europei di calcio del 2012, ma di sport, come diciamo noi, allo stato puro non riusciamo a parlare. Presidente, come dicevo poco fa, Alleanza Nazionale si asterrà dalla votazione, fedele al principio che non si vota una delega a questo Governo. Il Gruppo di Alleanza Nazionale, con competenza ed umiltà, ha contribuito a migliorare un testo che ci auguriamo non venga svilito, venga svilito, non sia disatteso dal Governo nella fase di attuazione della delega. Speriamo cioè che il Governo non vanifichi il parziale ma positivo lavoro svolto dal Parlamento.

Signor Presidente, anche il Gruppo di Forza Italia si asterrà nel giudizio finale su questo provvedimento, confermando l'approccio che abbiamo ricercato nel dibattito in Commissione,

ad interpretare ancora più correttamente un concetto che a noi è parso chiaro fin dall'inizio e che volevamo diventasse un patrimonio comune, quello di evitare le restrizioni, gli approcci rigidi e radicali attorno alla questione della Voglio fare una premessa, perché nel dibattito di questa mattina mi pare che un collega abbia recuperato una osservazione che, a mio modo di vedere, non c'entra alcunché: l'abbiamo detto in Commissione e lo ribadiamo quest'oggi. Non c'entra alcunché il disegno di legge che discutiamo questa mattina sui diritti televisivi come risposta ai fatti recenti di Calciopoli, allo scandalo che in qualche modo ha provocato un terremoto nel mondo del calcio, perché la questione di Calciopoli è cosa diversa. Immaginare una relazione di causa ed effetto tra le due questioni, come abbiamo detto, è assolutamente infondato e assolutamente privo di qualsiasi giustificazione. Diciamo questo, perché ci è parso in qualche modo poi consequenziale a questo rilievo il fatto di avviare una sorta di processo alla televisione digitale in quanto tale, dimenticando viceversa gli effetti positivi che ha generato l'avvento del digitale nel nostro Paese nella misura in cui ha avvicinato ancora di più un folto pubblico che prima giudicava, per così dire, eccessivamente onerosa la disponibilità di vedere il calcio e che ora dispone

La prima è l'approccio alla questione della vendita collettiva dei diritti calcistici, introdotta con questa norma: l'abbiamo detto in Commissione e lo ribadiamo qui. È vero, il percorso in Commissione ha contribuito ad attutire, ad organizzare meglio, a scrivere in maniera più corretta questo punto, però non vi è dubbio che, come è stato ricordato da tanti colleghi, l'introduzione della contrattazione collettiva porrà inevitabilmente problemi sul versante della legislazione, ad esempio, comunitaria, perché - lo ricordiamo - proprio a quel livello ci sono stati i maggiori interventi per tentare di legiferare in maniera tale che si rispettassero comunque i vincoli posti dall'articolo 81 del trattato UE sulla libera contrattazione e sulla concorrenza.

perché anche su questo versante a noi pare che gli accenti ad una sorta di intervento dirigistico possano essere considerati validi, così come ha recentemente ricordato lo stesso presidente dell'*Antitrust*.

di questo miglioramento, rispetto al quale do atto alla Commissione di avere svolto un buon lavoro. I suggerimenti che hanno modificato la norma originaria riguardano l'esclusività della piattaforma, per evitare di creare pericolose situazioni di monopolio, specie per quanto riguarda il satellite, atteso che se non avessimo mitigato quella norma avremmo finito per fare un grandioso regalo È stato anche attenuato il divieto, che a noi è sembrato opportuno sottolineare e richiedere, riguardo alla sub-licenza tra le diverse piattaforme, che costituisce un elemento fondamentale per garantire un accesso agevole a tutti gli utilizzatori. Con l'accoglimento di queste proposte - voglio ribadirlo ai colleghi - non abbiamo guardato con interesse a un gruppo, non abbiamo favorito una società, non abbiamo guardato a tutelare gli interessi di chi opera nel settore televisivo: a mio modo di vedere abbiamo favorito i consumatori in quanto tali, per far sì che gli utenti possano accedere al prodotto calcio in maniera più semplice, in un regime di maggiore concorrenza. Concludo, signor Presidente, auspicando che il Governo, nell'esercizio della delega, sappia recepire e mantenere vivo questo clima di collaborazione che abbiamo instaurato nel dibattito in Commissione ed anche in Aula con norme assolutamente coerenti con quanto è stato detto questa mattina.

Signor Presidente, il Gruppo Ulivo, come già detto dai relatori Mazzarello e Scalera, sostiene con convinzione la delega al Governo per una nuova disciplina dei diritti televisivi dello sport e della vendita centralizzata di tali diritti. Sulla questione della legge-delega si è già abbondantemente discusso alla Camera e al Senato, sia nelle Commissioni di merito che in Aula, e si può quindi affermare che la volontà del Governo e dei relatori di recepire gli indirizzi del Parlamento abbia delineato un quadro di riferimento normativo che circoscrive e delimita l'intervento delegato, valorizzando il ruolo del Parlamento nel chiarire gli orientamenti cui il Governo dovrà attenersi nell'esercizio della delega. Nel merito della questione, vi sono aspetti che meritano una seria riflessione politica e culturale prima ancora che legislativa. A partire dalla seconda metà degli anni Novanta, degli anni Novanta, si è andata affermando nel Paese una specie di mistica del mercato e delle sue regole, alle quali sono state attribuite virtù taumaturgiche per ogni settore di attività. Anche lo sport non ha saputo sottrarsi a questa idea, che nello specifico si è rivelata un'idea sbagliata. La logica della ricerca esasperata del solo profitto ha prodotto una degenerazione dell'iniziativa economica privata ed ha perciò indotto il Parlamento ad intervenire per tutelare quel bene comune che è lo sport. Alcune vicende hanno sconcertato l'opinione pubblica, provocando una forte perdita di credibilità del mondo del calcio: non mi riferisco solo a Calciopoli, ma anche alle plusvalenze con cui alcune società hanno aggiustato conti, si sono quotate in borsa, hanno disinvoltamente monetizzato i loro *brand*. Valutare in borsa le quotazioni dei calciatori genera evidenti distorsioni, solleticando tentazioni illegali di procuratori e calciatori; valutare in borsa, invece, come avviene in Spagna o Gran Bretagna, i grandi patrimoni immobiliari, le proprietà degli stadi e la gestione del marchio della società, assicura quotazioni che non compromettono il valore dello sport. Il calcio professionistico ha assunto una dimensione economica che sarebbe grave sottovalutare. Impegna migliaia di addetti, intrattiene stretti legami con il sistema delle comunicazioni e con la Borsa. Ritengo perciò che un approccio rigoroso agli aspetti economici vada a tutto beneficio della politica sportiva nella positiva tensione a far coincidere successo economico e risultato sportivo, per la soddisfazione del cittadino consumatore. È assolutamente necessario introdurre regole certe, applicabili, che si possano verificare senza generare un sistema tortuoso di procedure e controlli. La rilevanza economica dei diritti televisivi è tale da incidere per circa il 65 per cento nel bilancio delle società ed è evidente che le vendite soggettive dei diritti televisivi alimentano squilibri tra le società forti e quelle deboli. Per completezza di informazione e di analisi, ricordiamo che in Francia la vendita dei diritti televisivi è centralizzata, come lo è in Germania e in Inghilterra, sebbene con modalità tra loro diverse. Appare naturale quindi definire il disegno di legge in esame come una iniziativa opportuna, utile per introdurre elementi di rinnovamento in un sistema sofferente, attraverso la ridistribuzione e la mutualità. Per far ciò, tutte le piattaforme devono essere messe in condizione di contendersi i diritti: non tutti quindi nelle stesse mani, non tutti nella stessa piattaforma; tutti sotto l'attento esame e la puntuale vigilanza delle Autorità indipendenti di antitrust e di comunicazione. Durante i lavori in Commissione - come è stato ampiamente riferito - le problematiche inerenti la contabilità, la salvaguardia delle emittenti locali, la destinazione di quote ai fini di mutualità sono state ampiamente approfondite e su molte questioni si è trovato un comune terreno di intervento grazie alla disponibilità dei relatori e del Governo. Ne è emerso un disegno di legge che accentua, rispetto a quello della Camera, un'ampia intesa su questioni rilevanti.

soluzioni. Oggi si compie un passo significativo in tale direzione e perciò esprimiamo la nostra disponibilità al dialogo e il nostro voto favorevole.

Le forze dell'ordine, comandate dal vice questore Maione, hanno violentemente aggredito il Sindaco di quella cittadina, il presidente del Consiglio comunale, la vice Sindaco ed altri membri della popolazione. La ragione è che il commissario Bertolaso aveva provveduto a requisire il depuratore in costruzione a Nocera Superiore, Superiore, quindi non ancora collaudato per utilizzare le vasche - anche esse, lo sottolineo, non ancora collaudate - per sversare moltissimi camion provenienti da Villaricca con il percolato.

Poiché l'amministrazione del sindaco Montalbano è di centro-destra e il vice questore Maione è notoriamente legato ad un partito politico della maggioranza, credo che il Ministro dell'interno debba rispondere in ordine a questo fatto gravissimo.

chiedere alla Presidenza, se lo ritiene opportuno, di sollecitare un'informativa da parte del Governo. Tutte le altre affermazioni, legate anche all'attribuzione di collegamenti politici, mi sembrano gratuite e assolutamente da contestare. Peril resto, è evidente che su un episodio del genere occorre fare chiarezza. Ecco perché confido nella Presidenza affinché solleciti un intervento di chiarimento da parte del Governo, fermo restando che il collega potrà, con gli strumenti tipici del sindacato ispettivo, sollecitare una risposta anche in termini rapidi.

sulla domanda di autorizzazione a procedere in giudizio, ai sensi dell'articolo 96 della Costituzione, nei confronti del professor Antonio Marzano nella sua qualità di ministro delle attività produttive* pro tempore*, nonché dei signori Giovanni Bruno,

parlamentari ha proposto all'Assemblea di negare l'autorizzazione a procedere nei confronti del professor Antonio Marzano, nella sua qualità di Ministro delle attività produttive *pro tempore*, nonché degli altri coindagati. L'Assemblea delibererà separatamente su ciascuna di tali proposte di diniego. Tali proposte, in base al comma 8 dello stesso articolo 135-*bis* del Regolamento, s'intenderanno respinte qualora non conseguano il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti dell'Assemblea, cioè 162 voti. Come previsto dal comma 8-*bis* del medesimo articolo 135-*bis*, nella seduta antimeridiana avranno luogo la discussione e distinte votazioni nominali con scrutinio simultaneo. Di tali votazioni non verrà proclamato immediatamente il risultato. Successivamente, i senatori che non abbiano partecipato alle votazioni potranno recarsi sul banco della Presidenza e dichiarare il proprio voto ai senatori segretari. Tale facoltà potrà essere esercitata fino al termine della seduta antimeridiana e nel corso di quella pomeridiana fino alle ore 19, fatti salvi eventuali adeguamenti. Concluse le operazioni di voto, si procederà alle operazioni di scrutinio. Passiamo pertanto alla discussione del documento IV-*bis*, n.1-*bis*. Chiedo al relatore, senatore Manzione, se intende integrare la relazione scritta. Signor Presidente, il 3 novembre 2006 il Collegio per i reati ministeriali presso il tribunale di Roma ha nuovamente presentato richiesta di autorizzazione a procedere, ai sensi dell'articolo 96 della Costituzione, nei confronti del professor Antonio Marzano nella qualità, allora rivestita, di Ministro delle attività produttive nonché nei confronti di altri indagati, tutti per il reato previsto e punito dall'articolo 323, secondo comma, del codice penale, e cioè per abuso di ufficio, in relazione a vicende concernenti la nomina degli amministratori giudiziali nella procedura di amministrazione straordinaria per il gruppo ELDO S.p.A. Sulla precedente richiesta, nella seduta antimeridiana del 21 settembre 2006, dopo un ampio dibattito, veniva ulteriormente ribadito che l'incompletezza del quadro istruttorio offerto dal Collegio per i reati ministeriali, da un lato, rendeva configurabile quale unico esito possibile un provvedimento di archiviazione, che non rientrava naturalmente nei poteri del Senato e, dall'altro, privava il Senato stesso di elementi di conoscenza ulteriori dei quali *a priori* non poteva escludersi la rilevanza ai fini della sussistenza delle circostanze esimenti previste dalla legge costituzionale. Nel corso di quella seduta, l'Assemblea del Senato, che quindi si è già pronunciata su questa vicenda, aveva approvato la proposta della Giunta di restituire gli atti all'autorità giudiziaria per ulteriori approfondimenti. Il Collegio per i reati ministeriali presso il tribunale di Roma ha, invece, nuovamente chiesto l'autorizzazione a procedere, ai sensi dell'articolo 96 della Costituzione, nei confronti del professor Marzano, nella sua qualità di Ministro delle attività produttive *pro* *tempore*, nonché degli altri coindagati. Nel motivare la reiterazione della richiesta di autorizzazione, il Collegio per i reati ministeriali, e su questo punto chiedo ai colleghi di prestare un minimo di attenzione, ritiene che dagli atti del procedimento emergano inconfutabili dati fondanti la prospettata ipotesi accusatoria e che gli stessi fossero già stati ampiamente evidenziati nel provvedimento in data 2 maggio 2006. Tralasciando gli aspetti di carattere esclusivamente formale, a pagina 16 della nuova relazione che accompagna la richiesta del tribunale dei Ministri presso il tribunale di Roma si legge: «Alla luce di tutte le emergenze istruttorie or ora ripercorse, deve univocamente ritenersi che la scelta operata dal Ministro Marzano nella nomina in questione sia stata orientata in favore dei soggetti segnalati anche dallo stesso imprenditore, invece che improntata ai criteri del rispetto del buon andamento della P.A.». Questo Questo è un brano preciso della relazione che accompagna la seconda richiesta del cosiddetto tribunale per i Ministri, mentre, a pagina 14 della relazione originaria, lo stesso periodo era così formulato: «Alla luce di tutte le emergenze istruttorie di cui si è detto, deve univocamente ritenersi che, pur mancando la prova diretta di un intervento dei privati sulla persona del Ministro Marzano...» quindi, pur mancando la prova si diceva nella prima relazione - «...la scelta operata da questi della nomina in questione non sia stata assolutamente improntata a criteri di stretta discrezionalità». Dal confronto tra le due versioni emerge pertanto che, inizialmente, il Collegio per i reati ministeriali ha ritenuto che, sulla base degli atti processuali, non fosse comunque possibile considerare provato un intervento diretto dei privati sul ministro Marzano, in grado quindi di condizionare la nomina in questione ai fini non istituzionali, mentre, evidentemente, il problema della mancanza di questi elementi è considerato superato nella nuova relazione. Le considerazioni sopra esposte pongono in luce l'evidente differenza qualitativa dei giudizi che vengono formulati nelle due relazioni - è questo il punto, colleghi sulla base di un materiale istruttorio che è rimasto assolutamente immutato in relazione ai medesimi fatti. La decisione assunta nella seduta antimeridiana nel 21 settembre 2006 dall'Assemblea del Senato di restituire all'autorità giudiziaria gli atti concernenti la richiesta di autorizzazione a procedere sulla base delle motivazioni contenute nella relazione della Giunta implicava, per l'autorità giudiziaria, la necessità di procedere a compimenti di atti di ulteriore indagine per pervenire così all'adozione di un provvedimento di archiviazione o ad una valutazione di probabile fondatezza della notizia di reato e quindi ad una nuova richiesta di autorizzazione a procedere, ovvero, ovvero, non condividendosi la decisione assunta dall'Assemblea del Senato, alla possibilità di sollevare conflitto di attribuzione nei confronti del Senato medesimo. Il Collegio per i reati ministeriali, invece, ha scelto una strada diversa, richiedendo nuovamente al Senato l'autorizzazione a procedere sulla base di una rilettura del medesimo materiale istruttorio che ha però stranamente indotto il Collegio per i reati ministeriali a conclusioni assolutamente diverse e, in alcuni casi, oggettivamente contraddittorie rispetto a quanto affermato nella precedente relazione. In questa prospettiva appare quindi evidente come le determinazioni assunte dal Collegio per i reati ministeriali, per le modalità e i contenuti contraddittori delle medesime, risultino difficilmente compatibili con il rispetto di quell'obbligo di leale collaborazione su cui la Corte costituzionale e il nostro Senato hanno concordemente richiamato l'attenzione. In proposito, la Giunta, da un lato, ha preso atto della indisponibilità del Collegio per i reati ministeriali a prestare la collaborazione dovuta e, dall'altro, ha dovuto considerare l'opportunità di evitare, fin dove possibile, scelte che, dal punto di vista istituzionale, si sarebbero risolte in una vera e propria contrapposizione tra poteri dello Stato, quando risulta comunque possibile pervenire ad una valutazione positiva circa la sussistenza, signor Presidente, di almeno una di quelle due finalità che vengono indicate nell'articolo 9, comma 3, della legge costituzionale n. 1 del 1989. Più in particolare, nessun dubbio può esservi sul fatto che i risultati dell'azione del Ministro delle attività produttive *pro tempore* abbiano corrisposto alla realizzazione di un interesse pubblico nell'esercizio della funzione di Governo, interesse concretizzatosi nell'esigenza di tutelare le potenzialità del sistema produttivo ed i livelli occupazionali con specifico riferimento alla situazione del cosiddetto gruppo ELDO S.p.A. Ancora di più questa considerazione deve essere essere ritenuta pregnante ed incontestabile se si pensa che non siamo al cospetto di una nomina discrezionale da parte del Ministro, ma di un'indicazione obbligatoria che proveniva da una procedura che espressamente prevedeva quella competenza in capo al Ministro La valutazione complessiva degli elementi a disposizione della Giunta consente pertanto di pervenire ad una ricostruzione dei fatti nella quale l'azione del Ministro *pro tempore* per le attività produttive risulta contraddistinta, da un lato, dalla sua efficacia rispetto alle finalità di interesse pubblico ad essa sottese e, dall'altro, per l'assenza dei più significativi profili di anomalia segnalati dal Collegio per i reati ministeriali. Ciò non significa ovviamente escludere che la nomina dei commissari giudiziali nell'ambito della procedura ELDO S.p.A sia stata preceduta da iniziative di vario genere volte a far ricadere la scelta su alcune persone specificatamente specificatamente individuate. La Giunta, però, può senz'altro escludere che segnalazioni, raccomandazioni ed iniziative analoghe abbiano, nel caso di specie, condizionato la condotta del Ministro nell'esercizio delle sue funzioni, orientandola verso finalità diverse dallo specifico interesse pubblico che le deve essere sotteso alla luce del quadro normativo di riferimento. Milita a favore della considerazione di quest'ultima affermazione il fatto che lo stesso tribunale per i Ministri abbia più volte ripetuto nella prima relazione che mancava in maniera assoluta la prova diretta di un intervento e quindi di un collegamento dei privati con il ministro Marzano. Le considerazioni svolte hanno conclusivamente indotto la Giunta a ritenere che nella vicenda considerata il Ministro *pro tempore* per le attività produttive, professore Antonio Marzano, ha agito per il perseguimento di un interesse pubblico nell'esercizio della funzione di Governo e che tale interesse riveste senz'altro carattere preminente rispetto ad alcuni teorici profili di illegittimità, astrattamente ipotizzabili sulla base peraltro di una ricostruzione dei fatti che, per le ragioni sovra esposte, non ha potuto non discostarsi, in alcuni casi in modo anche rilevante, da quella fatta propria dal Collegio per i reati ministeriali. Ecco perché, Presidente, la la Giunta ha proposto di negare l'autorizzazione a procedere nei confronti del professor Antonio Marzano e degli altri coindagati. Tali conclusioni, a nome della Giunta, rivolgo all'Assemblea, chiedendo espressamente che il Senato neghi

Presidente, onorevoli colleghi, intervengo per conto del Gruppo dell'Ulivo per motivare il parere positivo alla proposta qui avanzata dal relatore, senatore Manzione, a nome della Giunta, proposta - come abbiamo sentito - di negare l'autorizzazione a procedere nei confronti del professore Antonio Marzano, già Ministro delle attività produttive, e di altri in merito al reato contenuto nella richiesta del Collegio per i reati ministeriali

Le vicende riguardano appunto la nomina degli amministratori giudiziali del gruppo ELDO S.p.A e della società ELDO S.p.A in amministrazione straordinaria. Ricordo ancora a tutti noi che la storia di questo procedimento vede una prima fase istruttoria che si conclude con una disposizione da parte del tribunale dei Ministri di archiviazione ed una successiva, sulla base di indagini ulteriori legate pertanto ad altri fatti in qualche modo connessi, che diversamente giunge alla richiesta di concessione della autorizzazione a procedere, ai sensi dell'articolo 96 della Costituzione, nei confronti dell'allora ministro Marzano. Il Collegio per i reati ministeriali presso il tribunale di Roma, pur escludendo ipotesi di reato più grave come - per esempio - la corruzione, ritiene che l'individuazione dei professionisti nominati in qualità di commissari giudiziali sia stata ispirata a criteri di favore e non invece a criteri di imparzialità, ed inoltre che le scelte siano state in qualche modo manipolate, comunque pilotate, da altri e non compiute secondo la piena discrezione secondo le prerogative del Ministro. In definitiva, essendo queste nomine finalizzate ad interessi di tipo privatistico, che ci sia stata una evidente violazione dell'articolo 323 Vorrei evidenziare che è lo stesso Collegio a sottolineare come il tribunale per i reati ministeriali abbia contemporaneamente compiti sia d'indagine che di giudizio. Pertanto, la richiesta di autorizzazione a procedere sarebbe, secondo il Collegio, l'unica alternativa alla procedura di archiviazione, procedura che sarebbe possibile solo in presenza di elementi di palese infondatezza.

con lo scopo di provocare un pronunciamento più esplicito da parte del Collegio. Ho voluto richiamare succintamente i fatti per contestualizzare la motivazione

secondo la legge possiamo, a maggioranza assoluta, negare l'autorizzazione a procedere, lì dove si reputi che l'inquisito, in questo caso l'ex ministro Marzano, abbia agito per la tutela di un interesse dello Stato, un interesse costituzionalmente rilevante, ovvero abbia agito per il perseguimento di un preminente interesse pubblico nell'esercizio della funzione di Governo.

non è sostenuta da ulteriori elementi di prova e da indagini suppletive e che, in più occasioni, lascia emergere valutazioni ed affermazioni contraddittorie con la precedente relazione. Appare pertanto fondata e condivisibile la lettura del relatore che è quella dell'insufficienza, dell'incompletezza e della non univocità delle risultanze: una valutazione che non consente a quest'Assemblea di fare proprie le conclusioni cui perviene il Collegio e, comunque, certamente non in maniera inequivocabile e incontrovertibile,

particolare, il fatto che il professor Marzano abbia voluto porre l'accento sulle molte altre situazioni di crisi aziendale e finanziaria

o contestazioni di illegalità nelle nomine, ma anzi, al contrario, come la sua bussola in questo, come in tutti gli altri casi, sia orientata nel senso di porre la massima attenzione alle aziende, alla necessità del loro risanamento finanziario e produttivo e, insieme, alla tutela di migliaia di lavoratori e di famiglie interessate (in questo caso parliamo di 250 lavoratori), mettendo chiaramente in luce un'ispirazione netta in direzione del perseguimento di obiettivi d'interesse sociale e, quindi, di finalità pubbliche e di rispetto delle leggi. A questo proposito, più volte lo stesso Marzano ha sottolineato, peraltro, come il suo operato si sviluppasse in assenza di un Regolamento sulle stesse nomine, Regolamento più volte

di avere regolamenti più chiari per quanto riguarda le nomine. Su questo argomento, tra l'altro, io e altre senatrici abbiamo presentato un progetto di legge.

per l'assenza di regole: in questo caso, ci auguriamo che le regole siano conseguenti anche alla nostra Costituzione e che diano trasparenza effettiva al sistema delle nomine. Spero che faremo tesoro anche di questa esperienza. Per tutte queste ragioni,

in quanto i senatori che non abbiano potuto partecipare ai voti elettronici potranno comunicare il voto ai senatori segretari, che ne prenderanno nota in apposito verbale. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, sulle conclusioni della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari volte a negare la concessione dell'autorizzazione a procedere nei confronti del professor Antonio Marzano, nella sua qualità di ministro delle attività produttive *pro tempore*. I senatori che, concordando con la proposta della Giunta, intendono negare l'autorizzazione a procedere, voteranno sì. I senatori contrari alla proposta della Giunta voteranno no. I senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza. Dichiaro aperta la votazione.

Non abbiamo, ovviamente, la proclamazione del risultato. **Votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, sulle conclusioni della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari volte a negare la concessione dell'autorizzazione a procedere nei confronti di Roberto Marraffa. Dichiaro aperta la votazione.

e delle immunità parlamentari volte a negare la concessione dell'autorizzazione a procedere nei confronti di Carlo Lancella. Dichiaro aperta la votazione.

la concessione dell'autorizzazione a procedere nei confronti di Carlo Lancella. Dichiaro aperta la votazione.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, sulle conclusioni della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari volte a negare la concessione dell'autorizzazione a procedere nei confronti di Carlo Lancella. Dichiaro aperta la votazione.

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, sulle conclusioni della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari volte a negare la concessione dell'autorizzazione a procedere nei confronti di Ernesto Marzano. Dichiaro aperta la votazione.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, sulle conclusioni della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari volte a negare la concessione dell'autorizzazione a procedere nei confronti di Walter Cretella Lombardo. Dichiaro aperta la votazione.

volte a negare la concessione dell'autorizzazione a procedere nei confronti di Ernesto Marzano. Dichiaro aperta la votazione. *(Segue la votazione).*

credo che l'andamento dei nostri lavori potrebbe portare - ovviamente se c'è la vostra collaborazione fattiva - all'esame

Questo emendamento, per l'appunto, riguarda le intercettazioni telefoniche. Con esso si vuole affermare che le intercettazioni che che non vengono acquisite dal giudice per le indagini preliminari al processo penale non possono essere utilizzate nel procedimento disciplinare. Che cosa significa ciò? La nostra Costituzione consente le intercettazioni telefoniche dietro provvedimento motivato dell'autorità giudiziaria e con riferimento esclusivamente a talune tipologie di reati; ad esempio, tutti i reati per i quali è prevista una pena non inferiore nel massimo ad anni cinque non possono essere oggetto di intercettazioni telefoniche. Queste ultime quindi servono per corrispondere alle esigenze dell'interesse punitivo dello Stato con riferimento a reati di particolare gravità. Non solo, ma il nostro ordinamento prevede che quando nel corso di un'intercettazione telefonica emergono elementi, per così dire, indizianti con riferimento a un reato diverso da quello per cui l'intercettazione è stata disposta, le intercettazioni possono essere utilizzate in altro procedimento solo se per il reato è previsto l'arresto obbligatorio, cioè per reati di particolarissima gravità. Orbene, se la norma di cui all'emendamento non dovesse entrare in vigore si verificherebbe, come si verifica normalmente, quanto segue. è la seguente: nel corso delle intercettazioni telefoniche emerge, ad esempio, che il dipendente pubblico "A" e la dipendente pubblica "B" hanno dei convegni amorosi all'interno del loro ufficio, circostanza che potrebbe, per ipotesi, assumere un rilievo disciplinare. Tale intercettazione, destinata nel processo penale a restare segreta, e che oggettivamente non è sostenuta, proprio per la sua irrilevanza penale, dalla necessità dell'intercettazione, viene veicolata nel procedimento disciplinare, diventa pubblica ed è alla base di un eventuale procedimento disciplinare. La seconda circostanza da un'intercettazione telefonica emerge che il dipendente pubblico ha commesso un determinato reato, diverso da quello per cui si intercetta. Orbene, siccome questo reato non prevede l'arresto obbligatorio, quella intercettazione non può essere utilizzata in fase processuale penale, per cui verrebbe veicolata solo nel procedimento disciplinare. In ordine a quella intercettazione vi sarebbe la risposta del dipendente pubblico e la risposta del dipendente pubblico veicolerebbe l'intercettazione nel processo penale,

che ha introdotto novità in forza delle quali sia la sentenza penale irrevocabile di condanna sia la sentenza di applicazione della pena su richiesta (il cosiddetto patteggiamento) sono destinate ad esplicare effetti nel giudizio disciplinare: questa è la correlazione fra

è una contrarietà da parte mia anche rispetto all'articolo 3, che per quanto riguarda l'ipotesi di decadenza del procedimento disciplinare prevede l'obbligo della

trasforma la comunicazione da parte dell'amministrazione giudiziaria nella ricezione della sentenza da parte dell'ufficio competente ad avviare il procedimento disciplinare. Questo significa che un termine di decadenza che doveva essere collegato ad un momento

assolutamente indeterminabile. Infatti, parlare di ricezione da parte dell'ufficio che deve promuovere non significa comunicazione all'amministrazione, ma comunicazione all'amministrazione da parte dell'autorità giudiziaria, stabilire quale ufficio deve promuovere l'azione disciplinare e quant'altro. Si è reso, quindi, questo termine assolutamente indeterminabile, e non sono d'accordo. Per venire all'emendamento in

che nei procedimenti disciplinari nei confronti di pubblici dipendenti non possano essere utilizzate quelle intercettazioni che non abbiano ricevuto il vaglio previsto dall'articolo 268, comma 6, del codice di procedura penale. Ciò significa

prima che terminasse la fase delle indagini preliminari e avvenisse il vaglio da parte del GIP. Si può verificare che quelle intercettazioni, immediatamente utilizzate nel procedimento disciplinare, vengano invece caducate dal provvedimento del GIP, che sottopone a verifica l'attività del pubblico ministero. In questo modo, invece, consentiamo che intercettazioni eventualmente illegittime fatte dal pubblico ministero

il provvedimento che regola le intercettazioni anche sotto il profilo della tutela della *privacy*. Dobbiamo renderci conto che in questo modo non solo corriamo il rischio di far transitare nel procedimento disciplinare

Ecco perché condivido sotto tutti i profili l'emendamento che il collega Palma ha presentato. Mi permetto di rivolgermi al relatore, alla sua grande saggezza, alla sua capacità di leggere anche in filigrana i provvedimenti, per chiedergli

oggetto dell'emendamento non ha attinenza con il provvedimento in questione. Sarebbe però una risposta sbagliata e soprattutto da non dare ai tre illustrissimi colleghi che l'hanno sottoscritta. Vorrei fare due osservazioni. La prima attiene alla natura del procedimento, sul quale bisogna riflettere. Il collega Manzione poco fa lo ha accennato: il procedimento penale è lo strumento nel quale si verifica la fondatezza dell'accusa e quindi massime devono essere le garanzie nei confronti dell'inquisito; nel procedimento disciplinare, invece, si deve verificare la possibile permanenza dell'incolpato nel posto di lavoro. Le garanzie debbono esserci, tuttavia diversa è la finalità, perché diverso è lo strumento da utilizzare. Credo che tutti possano cogliere la differenza che passa tra il delitto e la colpa: l'incolpato risponde di fronte all'ente circa la permanenza nel posto di lavoro, l'imputato risponde invece davanti al giudice circa la sussistenza di elementi tali da poterlo o meno condannare. dico che nel processo disciplinare vengono meno le garanzie, certamente però la finalità del procedimento disciplinare è quella di tutelare l'ente, lo Stato, l'azienda per il fatto che quel personaggio, pur essendo innocente rispetto al reato a lui addebitato, ha tuttavia delle colpe, per cui occorre verificare se può rimanere nel posto di lavoro.

di finanza furono imputati di corruzione e poi addirittura di concussione. La prova era così evidente che giustamente i difensori consigliarono loro di patteggiare la pena. La pena fu patteggiata quei due alti ufficiali tornarono negli stessi posti che rivestivano quando commisero i reati di corruzione e concussione. Questo non possiamo consentirlo. Lo voglio ricordare per la necessità di approvare questa legge, ma nello stesso tempo per ricordare la differenza che vi è tra delitto e colpa. Anche questo è un argomento non sufficiente a dirimere il problema: lo so bene.

è una corposa norma di riforma e di modifica dell'articolo 268 del codice di procedura penale

abrogati». Ci troviamo allora di fronte a due norme: da una parte una legge concernente l'utilizzabilità delle intercettazioni nel processo disciplinare che riguarda la nostra legge

Manzione, mi consentirà di osservare che si tratta di due norme in aperto conflitto, in questo momento. Se approviamo una norma che prevede l'utilizzabilità del comma 6 dell'articolo 286, avremo di fronte, poi, la decisione rispetto ad una legge, quella sulle intercettazioni, nella quale questa norma viene abrogata. tratta di una norma che certamente merita attenzione e interesse, non va sottovalutata e trattata come se fosse una questione

Qual è la soluzione che propongo? Siccome la Camera dei deputati ha approvato, pressoché all'unanimità, l'abrogazione del comma 6 dell'articolo 286, piuttosto che richiamarlo in questa sede

dobbiamo assolutamente evitare che si crei un conflitto del genere tra due leggi, è vero, ambedue non approvate, ma se approvassimo in questa sede...

Ricordo che il provvedimento non riguarda il procedimento disciplinare, ma i rapporti tra il procedimento penale e il procedimento disciplinare, e intende sanare un fenomeno molto grave a parere di tutti, cioè che troppi condannati per la durata del procedimento e per i nessi difficili e burocratici tra procedimento penale e procedimento disciplinare rimangono al loro posto di lavoro con lo stesso ruolo che ha consentito loro di gravi di concussione, corruzione e peculato contro la pubblica amministrazione. Ricordo inoltre - come ha già fatto il relatore - che la materia delle intercettazioni è già oggetto di una ulteriore iniziativa legislativa all'esame della Camera